con le quali le onorevoli senatrici chiedono notizie riguardo all'emanazione del decreto che autorizza le scuole secondarie di primo grado statali "Rinascita A. Livi" di Milano, "Don Milani-Colombo" di Genova e "Scuola-Città Pestalozzi" di Firenze ad attuare il progetto sperimentale elaborato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Al riguardo, il ministro Gelmini, in data 14 giugno 2011, ha firmato il decreto con il quale viene autorizzata, con decorrenza 1° settembre 2011, la sperimentazione del progetto predisposto dalle scuole citate. Detto progetto sperimentale prevede una rete di istituzioni scolastiche attraverso la quale l'attività di ricerca innovativa possa coerentemente integrarsi con gli interventi di carattere didattico-pedagogico e organizzativo legati alla concreta applicazione della riforma di cui al decreto legislativo n. 59 del 2004, che ha definito le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, anche in relazione alle indicazioni provenienti da esperienze internazionali. Le istituzioni scolastiche partecipanti alla rete assumono altresì la funzione di scuola laboratorio per la ricerca, sperimentazione e diffusione sul territorio di soluzioni applicative, anche mediante la costituzione di ulteriori reti locali. relativo alla formazione, prevede il consolidamento e lo sviluppo dei «Centri risorse per la formazione professionale dei docenti» delle scuole del territorio, già avviato con decreto ministeriale del 10 marzo 2006. Il piano didattico-organizzativo comprende lo studio e la sperimentazione di soluzioni applicative relative alle innovazioni di sistema. La complessità del progetto richiede la partecipazione di personale fortemente motivato, che sia disponibile a condividere le esperienze della sperimentazione ed innovazione di sistema con i docenti in servizio in altre scuole. Il progetto valorizza l'autonomia delle scuole interessate, rimettendo alle loro determinazioni le modalità di coordinamento del medesimo e di rendicontazione verso l'amministrazione centrale. Per lo svolgimento delle attività integrate specifiche è assegnato un organico funzionale sperimentale finalizzato a garantire l'attività di insegnamento, di formazione, di ricerca didattica e di documentazione. La sperimentazione avrà durata biennale e potrà essere, eventualmente, rinnovata.

elusione. Queste scuole, infatti, avevano in scadenza un progetto triennale e hanno presentato - come richiesto - un nuovo progetto triennale; se non sono male informata, il decreto cui lei ha fatto riferimento

Rinascita, che nasce sulla spinta delle volontà locali: una scuola nata dal basso. Essa aveva prima uno statuto di tipo privatistico; poi è entrata giustamente nel sistema scolastico nazionale,

rappresentano un modello a rete (che dovrebbe essere alternativo al modello centralistico e burocratico calato dall'alto), basato sull'autonomia (altro tema che dovrebbe essere connesso ad una visione federalista

per permettere a queste scuole - che, come il Sottosegretario ha detto, sperimentano per poter diffondere, perché mettono insieme ricerca, formazione e rete - di continuare a a svolgere la loro funzione, al servizio non solo dei loro territori che le hanno volute, e che ancora le difendono, ma di tutta le scuola italiana. [FRANCO

soddisfatta, nel senso che finalmente, sia pur con ritardo, questa risposta del Ministero è poi arrivata ed è stata positiva;

sinceramente è davvero un periodo troppo breve per poter attuare una sperimentazione della portata di quella indicata nel progetto

2006-2011, riguardava un periodo di cinque anni. Cinque anni sono un periodo congruo per poter realizzare e valutare la portata e gli effetti

mira a sviluppare - dicono i presentatori - un modello di scuola che risponda meglio ai bisogni degli studenti nell'era digitale. Mi sembra un bellissimo progetto, che potrebbe portare la la qualità della didattica nel nostro Paese ad un livello davvero alto e più rispondente alla cultura e all'essere dei giovani studenti oggi. oggi. Due anni sinceramente sono davvero pochi, soprattutto se c'è la spada di Damocle della proroga, che potrebbe esserci o meno. Tutto questo rende più precario il lavoro di ricerca, e lei sa benissimo che la ricerca realizzata in condizioni di precarietà parte già male.

e innovazione che possono essere utili anche per la formazione degli insegnanti. È un elemento di qualità che il Ministero dovrebbe valutare, considerando queste scuole un'opportunità e non un costo.

a causa della presenza di un numero di iscrizioni di cittadini stranieri superiore al 30 per cento. Al riguardo, si premette che la presenza nelle scuole di alunni di diversa provenienza geografica a cui si accompagnano una differente formazione culturale ed esperienze di apprendimento, costituisce oramai un dato strutturale in continuo aumento. Questo generalizzato e complesso fenomeno presenta aspetti problematici e criticità, che comunque non fanno venir meno l'obiettivo prioritario del sistema scolastico nazionale di favorire per tutti gli studenti la crescita delle delle capacità autonome di studio ed apprendimento ed il rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale. Ciò comporta la necessità di coniugare efficacemente la massima inclusione degli studenti di cittadinanza non italiana con un'offerta formativa qualitativamente valida, che tenga conto delle situazioni di partenza e delle esigenze di ciascun alunno. La molteplicità di culture ed esperienze non può tradursi in condizioni di disagio e di difficoltà che portano all'insuccesso scolastico, all'abbandono ed al ritardo nei percorsi di studio, ma rappresenta uno stimolo all'adozione di modalità organizzative e di metodologie didattiche adeguate alle nuove esigenze, che contribuiscono a creare l'indispensabile condivisione delle norme della convivenza e della partecipazione sociale. Sul piano organizzativo è indubbio che la presenza nelle classi di alunni con livelli di scolarizzazione fortemente disomogenei presenta un oggettivo fattore di rischio di parziale o totale insuccesso formativo per gli alunni coinvolti. Costituisce in sostanza una criticità che si riverbera sul complessivo processo di apprendimento dell'intera classe. L'effettiva integrazione di alunni con cittadinanza non italiana rappresenta allora una necessità ineludibile e non un astratto intento. A tal fine una buona conoscenza della lingua italiana è un requisito indispensabile per il buon esito del percorso scolastico e di un armonioso inserimento sociale, il cui conseguimento partecipa anche della condivisione dei principi di legalità e di democrazia. È noto in proposito che l'apprendimento della lingua, soprattutto tra i giovani, migliori con l'aumentare dell'esposizione scolastica e con l'uso quotidiano nell'ambiente scolastico. È pertanto preferibile stimolare lo scambio di opinioni tra studenti di diversa provenienza, evitando la formazione di gruppi autonomi ed a se stanti che anche in ambiente scolastico utilizzano la lingua originaria. In questa prospettiva il Ministero ha adottato alcune nuove e finalizzate misure organizzative che integrano le iniziative già sperimentate con successo sul territorio. Le misure in oggetto, attraverso una attenta analisi della situazione specifica dei singoli contesti, valorizzano l'inclusione equilibrata ed efficace di alunni stranieri, in grado di favorire il positivo sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento sia per l'istituzione scolastica nel suo complesso, sia per tutti i singoli alunni e studenti. La procedura prevede la programmazione del flusso delle iscrizioni con azioni concertate con l'ente locale e la prefettura e gestite in modo strategico dall'ufficio scolastico regionale. La definizione delle condizioni per assicurare a tutti opportunità di istruzione è connessa con la fissazione di limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana. Per questi motivi il numero di alunni di cittadinanza non italiana presenti in ogni classe non può superare di norma il 30 per cento del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana che insistono sullo stesso territorio. Il limite fissato è introdotto in modo graduale a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e può essere innalzato, con determinazione del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, in caso di presenza di alunni stranieri in possesso di adeguate competenze linguistiche. Di contro, il suddetto limite può essere abbassato dallo stesso direttore a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti all'atto dell'iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata per la compiuta partecipazione all'attività didattica e comunque a fronte di particolari e Al buon esito della procedura devono tendere in modo sinergico, ognuna per la parte di competenza, tutte le istituzioni interessate, uffici scolastici regionali e territoriali, prefetture, province, comuni, istituzioni scolastiche, attraverso la costruzione di veri e propri patti territoriali, che consentano un'equilibrata gestione dei loro bacini di utenza. È così possibile anno per anno gestire nel modo ottimale i flussi delle iscrizioni attraverso l'indizione di conferenze di servizio e la previsione di modalità di governo coordinato della quota eccedente il 30 per cento della singola scuola. Gli stessi criteri organizzativi si applicano nella composizione della singola classe. L'inserimento nelle classi degli studenti di cittadinanza non italiana è accompagnato dall'adozione di una serie di misure e iniziative che favoriscono la loro effettiva integrazione e assicurano un efficace processo di insegnamento-apprendimento. Mi riferisco in particolare all'attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana di gruppi di livello, sia in orario curricolare sia in corsi extracurricolari; all'utilizzo della quota di flessibilità del 20 per cento per corsi di lingua italiana di diverso livello; alla partecipazione a progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua; all'inserimento scolastico degli alunni stranieri neoarrivati in corso d'anno attraverso la partecipazione ad attività finalizzate ad acquisire un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, anche mediante corsi intensivi propedeutici, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica. In questo contesto alle scuole, anche con la mediazione del privato sociale, è assegnato un ruolo di stimolo all'organizzazione di situazioni relazionali e di socializzazione tra coetanei in ambito extracurricolare che favoriscono l'uso della lingua italiana. La messa in opera dei nuovi criteri richiede da parte di tutti i soggetti coinvolti una gestione attenta, coordinata, puntuale ed esente da ogni rigidità burocratica. Il limite del 30 per cento deve essere modulato e calibrato in rapporto al singolo contesto territoriale ed alle dimensioni e caratteristiche del fenomeno migratorio. Detto limite può essere superato in presenza di studenti che abbiano un'adeguata competenza della lingua italiana; qualora vi siano risorse professionali e strutture di supporto, anche esterne alla scuola, in grado di contribuire fattivamente al processo di apprendimento, o vi siano ragioni di continuità didattica di classi già costituite negli anni precedenti; in presenza, infine, di stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative. È allora di tutta evidenza che sia privo di fondamento ricondurre la mancata autorizzazione di una classe aggiuntiva, rispetto alla singola prevista, alla scuola serale per lavoratori per il fatto che oltre il 30 per cento degli iscritti sia di cittadinanza straniera. Al riguardo l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia precisa che, come illustrato nel corso degli incontri di informativa alle organizzazioni sindacali regionali, in questa procedura non assume alcuna rilevanza che la percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana iscritti ai corsi serali dell'istituto sia superiore alla quota stabilita dalla circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010. Il risalto attribuito al caso da alcuni organi d'informazione ha indotto lo stesso direttore generale e il dirigente dell'ambito territoriale di Milano a pubblicare sui siti *web* dei rispettivi uffici appositi comunicati stampa, con i quali smentiscono che la mancata autorizzazione sia riconducibile al superamento del tetto del 30 per cento di alunni stranieri, non ritenendo detto limite immediatamente applicabile ai corsi serali. In realtà, è noto che il numero delle iscrizioni ai corsi serali subisce rilevanti variazioni che possono tradursi in una scarsa efficienza delle risorse assegnate. Per questi motivi l'ufficio regionale evidenzia come, in materia di corsi serali, la gestione dei posti attivabili in organico di diritto sulla base delle esigenze al momento accertate non sia attendibile e sia, al contrario, preferibile rinviare la valutazione sulla definitiva attivazione delle classi alla fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, potendo fare affidamento su dati certi di consistenza degli iscritti. Sono state così autorizzate in questa fase cinque classi aggiuntive rispetto a quanto previsto in organico di diritto, risultando ora funzionanti tre classi prime e due classi per ciascuno degli anni successivi del corso di studi. Preciso, infine, che la serie storica dei dati del corso serale in questione attesta la presenza di una forbice tra gli studenti iscritti e quelli effettivamente frequentanti, che tende ad ampliarsi subito dopo l'inizio dell'anno scolastico per attestarsi, al termine dell'anno, in una percentuale di studenti scrutinati che oscilla tra il 30 ed il 40 per cento degli iscritti.

lo ringrazio anche perché ha cercato di entrare nella lettura della situazione di un istituto professionale di Milano, il «Bertarelli», dei corsi serali in una città che ha una presenza e una frequenza crescente di ragazzi provenienti da altre culture. i vostri criteri, a mio parere, sono del tutto insufficienti per lavorare su una materia così complessa, ma anche così chiara.

il dirigente regionale deve avere rapporti con tutti i soggetti istituzionali e sociali e studiare con loro il modo per offrire opportunità formative.

l'organico funzionale è costituito da un numero di posti aggiuntivi, con la loro stabilità a disposizione della progettazione interna ad una realtà molto forte, magmatica ed in movimento, che non può essere imbrigliata dal criterio del 30

alla prova preselettiva del concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici ed iniziative per l'accertamento della responsabilità per la fuga di notizie. Al riguardo sono pervenute anche numerose segnalazioni di varie associazioni di categoria, tra cui quella dell'Associazione nazionale presidi ed una richiesta di notizie da parte della Polizia postale. Questo Ministero ha, pertanto, predisposto una dettagliata relazione con cui si ripercorre l'*iter* della consegna del cd-rom contenente il *file* dei *test* preparati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e della successiva lavorazione del *file* da parte dei tecnici informatici sino alla pubblicazione dello stesso in data 1° settembre 2011. Allo stato attuale non emergono prove e responsabilità fondate sulla presunta diffusione anticipata dei quesiti a risposta multipla che, comunque, non pregiudica la prosecuzione del concorso. L'intera procedura prevede il coinvolgimento ed il supporto dell'ANSAS e di Formez e si basa sulla trasparenza degli atti ed economicità di gestione. L'ANSAS ha curato la predisposizione del contenuto dei quesiti e la presenza di refusi e/o errori nella batteria dei *test* è comune a qualsiasi altra procedura concorsuale in cui vi sia la preventiva pubblicazione dei quesiti, la cui funzione è strettamente collegata all'esigenza di trasparenza e di rendere possibile la segnalazione di errori. Si tratta di una percentuale fisiologica di imprecisioni o refusi tale da non inficiare la qualità del lavoro svolto e delle domande pubblicate. Comunque, tutti i quesiti segnalati che contengono refusi o formulazioni ambigue, previo esame di un gruppo di lavoro appositamente costituito, saranno esclusi dal sorteggio finale garantendo così l'estrazione da una banca dati collaudata. Formez, invece, si occuperà della stampa del materiale di esame e della successiva correzione. L'adozione della procedura selettiva Ripam del Formez, assicura trasparenza ed economicità, è stata validata dalla commissione interministeriale e, recentemente, è stata positivamente analizzata anche dall'università «Bocconi». La procedura prevede la consegna ai candidati di un volume di carta riciclata contenente le domande inserite nella banca dati pubblicata dalla quale, il giorno della prova, saranno estratti a caso i 100 quesiti oggetto dell'esame. Fino a pochi istanti prima dell'inizio della prova, nessuno è a conoscenza dei quesiti sorteggiati. Il costo di ogni volume (circa 2 euro) è nettamente inferiore ai costi dei materiali, del personale, dell'affitto delle fotocopiatrici e di tutte le altre voci di spesa che sarebbero intervenute qualora non si fosse seguita questa procedura concorsuale. Il Ministero, d'altra parte, ha adottato le stesse modalità già sperimentate negli ultimi anni in occasione dello svolgimento dei concorsi per la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ISTAT.

non è una buona cosa. Si dice poi che sono avvenute con grande economicità, ma io aggiungo che l'insieme delle prime procedure in attuazione delle norme previste dal bando

- credo correttamente - che si tratta di una prova diretta all'accertamento del possesso delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale. Orbene, rispetto alle aree tematiche ivi indicate (che sono otto), nell'insieme - non so se li avete letti - sono una cosa pazzesca. Di fatto, il Ministero affida la selezione della dirigenza scolastica a criteri del tutto privi di senso, cioè al caso.

la formula in sé, macchinosa e nozionistica, di una prova di preselezione, al di là poi delle prove del concorso, che viene impiegata per la eliminazione reale di moltissimi concorrenti.

È una cosa gravissima, perché così si mina la qualità del sistema scolastico italiano circa gli esiti di una selezione di questo genere; in secondo luogo, si manca di rispetto verso le persone che vengono dal mondo della scuola.

Quale candidato supererà la prova? Bisogna pur chiederselo, alla fine. Questa preselezione è un macigno su un concorso più lineare che avrebbe dovuto essere quello di merito.

Questo meccanismo garantisce la imparzialità? È una domanda che pongo in quanto non ho ottenuto una risposta tranquillizzante. Un'ultima cosa.

C'è stata un'incapacità gestionale politico‑amministrativa. C'è stata improvvisazione e leggerezza, e quindi mancanza di credibilità dell'azione politica e amministrativa. Non ci venga a dire che agisce in questo modo tutta la pubblica amministrazione: non ci posso credere. Temo - ahimè - che già da inzio nascerà parecchio contenzioso, anche - ad esempio - per la differenziazione del calendario regionale delle prove,

un meccanismo uniforme senza scarti, senza errori, la base del concorso che vi ostinate a mandare avanti è molto fragile, e credo che metta in discussione la validità del concorso stesso. Vorrei dire al Ministro che non si governa e non si amministra così, rappresentando lo Stato.